delle votazioni per l'elezione di un componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e** **di un componente del consiglio di presidenza

e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

nel mio intervento di insediamento: un giovane che perse la vita, da innocente, colpito sotto casa, sotto gli occhi della madre, per un odio politico che sono certo tutti rigettiamo, da qualunque parte provenga, e che ci auguriamo non trovi mai spazio

Signor Presidente, sarò abbastanza veloce, perché già ieri ho proceduto con la relazione iniziale e questa - come lei sa - è un'appendice alla relazione di ieri. Quindi, ella dovrà probabilmente sospendere la seduta dopo questo mio breve intervento. Il mio intervento riguarda la seduta di Commissione che si è svolta questa mattina, che mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2023, sulla Nuova Relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché sugli atti allegati. In relazione al DEF 2023, mi riporto all'illustrazione già svolta nella seduta di ieri, atteso che il Governo ha precisato che tale Documento non ha subito variazioni rispetto a quello presentato alle Camere il 12 aprile scorso. Con riferimento all'annesso *bis*, la Nuova Relazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, è stata trasmessa dal Governo il 27 aprile scorso, a seguito dell'esito della votazione della Relazione annessa al Documento di economia e finanza 2023 presso la Camera dei deputati. Con la presentazione di questa nuova Relazione il Governo ribadisce la richiesta dell'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissato per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022, vale a dire il 4,5 per cento nel 2023 e il 3,7 per cento nel 2024, a fronte di una previsione tendenziale di indebitamento netto in rapporto al PIL e al 3,5 per cento nel 2024. Con la presente Relazione il Governo, nel confermare l'intenzione di utilizzare il margine di bilancio resosi disponibile per il 2023, che ammonta a 3,4 miliardi di euro, per la copertura di un provvedimento di prossima adozione volto a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti, prevede altresì, rispetto alla precedente Relazione, che le predette risorse siano destinate anche al sostegno delle famiglie con figli. Per quanto riguarda il 2024, è invece confermata la destinazione delle risorse disponibili, consistenti in 4,5 miliardi di euro, a interventi di riduzione della pressione fiscale.

la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del Documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla Nuova Relazione di cui all'articolo 6,

I testi sono in distribuzione.

La prossima seduta sarà dopo il 1° maggio e penso sia giusto che quest'Assemblea ricordi con un minuto di silenzio le vittime degli incidenti sul lavoro, che credo meritino un riconoscimento unanime.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, non mi appartiene nascondere la faccia sotto la sabbia e quindi, nonostante il Senato della Repubblica abbia fatto appieno il proprio dovere ieri nel votare le risoluzioni sullo scostamento di bilancio e sul DEF, non c'è nulla da minimizzare: ieri alla Camera la maggioranza non ha fatto una bella figura innanzi agli italiani. Ma mi si lasci dire che non l'ha fatta nemmeno l'opposizione, che ora si accinge a dare fuoco... *(Commenti).* State calmi. PRESIDENTE.Senatrice Biancofiore, ci penso io. Vi

spettacolarizzazione in diretta televisiva, gettando fango sul Parlamento in un crescendo "tafazzista" che si ripercuote sulla credibilità di tutti noi e delle istituzioni. E spiego perché. Ieri alla Camera è stato bocciato non il DEF, cioè il Documento di economia e finanza del Governo - come erroneamente si è semplificato anche su alcuni *media* - ma la Relazione relativa allo scostamento di bilancio, ovvero il documento che autorizzava il Governo a mettere oltre 3,4 miliardi di euro sul taglio del cuneo fiscale e per il varo del decreto lavoro, del quale tanto vi riempite la bocca. In sostanza, non è stato approvato un documento che autorizzava il Governo a fare un debito per tagliare le tasse sul lavoro; un documento, dunque, che in una Nazione seria... *(Commenti)*.

c'era e c'è l'interesse nazionale di milioni di lavoratori e imprese. Mi corre l'obbligo di precisare che ieri...

la civiltà di ascoltarla senza protestare. Prego, Senatrice Biancofiore, prego anche lei. Rilevo un po' di nervosismo.

Ciò premesso, nonostante questo assurdo incidente di percorso - sarà però di insegnamento, nell'importanza di dare centralità al Parlamento, al valore e al lavoro di ogni singolo parlamentare, per il futuro della maggioranza, con una più stretta cinghia di trasmissione tra Governo e maggioranza anche il viaggio di ieri del *premier* Meloni a Londra è stato un successo, con l'elogio da parte del *premier* britannico Sunak, ancora una volta sulla politica economica del primo ministro Meloni. Sunak ha testualmente detto: «Voglio elogiare la tua gestione molto attenta dell'economia italiana, cosa che ha portato stabilità in tempi di incertezza» per poi affrontare insieme il *dossier* sulla lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina, con assolute convergenze sul *modus operandi* - che vi piaccia o meno - del Governo Meloni. Le parole di Sunak - *last but not least*, come dicono gli inglesi - seguono quelle dell'editoriale del «The Washington Post» sul bilancio positivo dei primi sei mesi di Governo

tanto per citarne solo alcuni dei più famosi. L'analisi del «The Washington Post» prende in considerazione come parametro di successo, ancora una volta, come Sunak, la politica economica del Governo Meloni, evidenziando l'approccio serio, pragmatico e risoluto con cui è stata scritta la legge di bilancio,

nell'Indo-Pacifico; la condivisione dei valori della NATO; l'appoggio incondizionato all'Ucraina e la visione strategica del Piano Mattei, che il Continente africano necessita, passando per un "*fact act*" politico sui migranti, che è fondamentale. Certamente sarebbe meglio che una parte dell'Europa avesse evitato di zavorrare l'Italia con una sorta di reddito di stabilità, come quello varato ieri. Ma l'Italia della Meloni non strepita e non urla al complotto, anche se l'intervento di certe agenzie di *rating* qualche sospetto desta; però e argomenta in forza della convinzione di un Paese che, nelle difficoltà, ha sempre dimostrato di dare il meglio di sé. In merito alle agenzie di *rating*, mi impegno a presentare un disegno di legge di istituzione dell'Osservatorio sulle agenzie di valutazione del merito e del credito, di *rating* appunto, nonché di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività delle medesime agenzie. Da anni, infatti, i comportamenti delle agenzie di *rating*, che si esplicano tramite i voti sull'affidabilità e sulla solvibilità delle imprese e degli Stati che emettono titoli di debito, destano più di una perplessità. Basti prendere uno dei casi più clamorosi tra gli errori compiuti da queste agenzie, come quelle della Parmalat in Italia o di Enron negli Stati Uniti. Ai *bond* della società di Collecchio, come a quelli dell'americana Enron le agenzie di *rating* avevano accordato, fino al giorno del *default*, i voti di affabilità massima: alla Enron addirittura la tripla A. Dopo il collasso della Parmalat se la sono presa, di fatto, soltanto con le banche, che avevano emesso un debito, che era stato approvato appunto delle agenzie di *rating*. In questo contesto, il Documento di economia e finanza che discutiamo oggi e che detta la linea del prossimo programma di bilancio è dunque cruciale e ancora una volta dimostra quella serietà e quella competenza evidenziata dai media internazionali con cui il Governo Meloni - vi piaccia o meno - pur facendo i conti con le difficoltà e i vari fronti emergenziali aperti, intende

delle famiglie, in particolare per quelle numerose, e delle imprese, e le misure destinate a rilanciare gli investimenti e rafforzare la competitività del Paese. *(Applausi)*. Va peraltro evidenziato come il Governo nella fissazione e nell'attuazione degli obiettivi abbia proprio tenuto alta l'attenzione sulla sostenibilità dei conti pubblici, impegnandosi anche a una graduale riduzione del del *deficit* e del debito, in previsione anche della riforma del Patto di stabilità e crescita puntualmente varato l'altro ieri dalla Commissione europea, che ci consente flessibilità, ma ci richiede rigore nel rientro sul debito. Questa è serietà. Questo è perseguire l'interesse interesse nazionale e sono orgogliosa di far parte di questa maggioranza, che si dimostra responsabile rispettando gli impegni assunti *(Applausi)*, senza scaricare gli oneri sulle future generazioni. Dopo anni di oppressione fiscale, questo Governo segna la discontinuità e, invece che mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ha il coraggio di impiegare le maggiori risorse in via prioritaria nel taglio della tassazione. i segnali ci sono e sono positivi. In questi anni il sistema economico italiano si è dimostrato resiliente, rispondendo bene alle situazioni contingenti e reagendo meglio di molti *partner* europei con un debito inferiore al nostro. Secondo i dati di oggi di Eurostat - anche questo che vi piaccia o meno - l'Italia segna un + 0,1 per cento, risultando seconda in Europa per crescita. L'aumento delle previsioni per l'anno in corso è il nostro primo e importante risultato e ci consente di poter agire con più forte autorevolezza anche a livello comunitario. Questo nuovo clima di fiducia è attestato anche dalla significativa ripresa dei consumi delle famiglie. Dovremo cogliere tutte le opportunità che questo periodo ha portato con sé, in particolare proseguendo nella realizzazione di tutte le misure previste dal PNRR - come sostenuto dal ministro Fitto - che è un punto fondamentale non solo per l'ottenimento dei fondi, ma anche e soprattutto per la realizzazione delle riforme strutturali che il Paese da tempo aspetta. Abbiamo ancora qualche mese per lavorare sulla prossima legge di bilancio. Io voglio esprimere un auspicio nonostante il clima, ovvero che si superi questa voglia di divisione, questa balcanizzazione politica. Dobbiamo lavorare insieme nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, contribuendo però tutti a dare le risposte che gli italiani si aspettano. Per rilanciare il sistema Paese in modo duraturo sono fondamentali la coesione politica e la collaborazione più ampia possibile fra le istituzioni. Ad ogni modo ci tengo a rassicurare gli italiani che ci stanno ascoltando: questo Governo andrà avanti, proprio dopo questo incidente, con più forza, decisione e convinzione di quelle che l'hanno contraddistinto finora e che derivano da una legittimazione che gli elettori continuano ad accordarci in tutte le tornate elettorali, perché ci occupiamo dei problemi fondamentali delle persone, ci occupiamo veramente della povertà

voterà a favore di questo Documento nella consapevolezza che ci consentirà di gettare le basi per la crescita dei prossimi anni e di essere sempre dalla parte degli italiani e solo degli italiani.

Grazie, Presidente. uno scostamento di bilancio che - come ben sappiamo ormai - non ha ottenuto ieri alla Camera i voti necessari. Dico subito, all'inizio del mio intervento, che non ve la caverete certamente dicendo che è colpa degli altri. *(Applausi)*. Questo è però talmente evidente che non va nemmeno ribadito. È un inedito nella storia repubblicana, non era mai accaduto prima. Davvero complimenti. Non si tratta peraltro nemmeno di un incidente minore, un po' imbarazzante. Di fronte a uno scivolone così rovinoso è davvero inevitabile domandarsi quello che in questo momento si stanno certamente chiedendo milioni di italiani: se un Governo e una maggioranza non sono in grado nemmeno di completare l'obiettivo più semplice che si possa immaginare, quello cioè di portare in Aula i propri eletti, peraltro per un voto così importante, come potranno essere capaci di raggiungere obiettivi assai più difficili? Se il ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio è per il Governo troppo impervio, cosa succederà quando metterete mano al faraonico quanto inutile ponte sullo Stretto? Ma è solo imperizia? Forse no. Dietro questo brutto incidente - per citare le parole del *Premier* - ci sono in realtà anche le divisioni interne a questa maggioranza, molto più profonde di quanto non si voglia ammettere. Nonostante il potere sia un cemento assai possente, queste divisioni però stanno aumentando. Si era già visto una settimana fa con il decreto Cutro e si vede ancora di più adesso. Le divisioni non solo ci sono, ma diventa sempre più difficile nasconderle e negarle. Invece, a fronte delle crepe della maggioranza, consideriamo tutti noi molto positivo quanto fatto in questi giorni dall'opposizione o almeno da buona parte di essa. La risoluzione comune, firmata dall'Alleanza Verdi e Sinistra, dal Partito Democratico e dal MoVimento 5 Stelle, prova a disegnare un'idea di società. E questa unità ritrovata è un fatto - a mio avviso - molto importante, che certo non basta a sanare il gravissimo errore dell'estate scorsa, quando noi forze democratiche e progressiste ci siamo colpevolmente divise, spianando la strada alle destre, ma che va finalmente nella giusta direzione. Iniziamo a delineare insieme un progetto e una visione del Paese alternativi a quelli delle destre. Il vostro DEF non solo non ha una strategia e un'ambizione, ma ancora una volta penalizza i più deboli e aumenta le diseguaglianze sociali, invece di correggerle. *(Applausi)*. Come sempre vi comportate come una destra liberista, che non ha nulla di sociale. Eppure, la fiammata inflazionistica, che ha fatto crollare il potere di acquisto dei salari, avrebbe meritato una risposta assai diversa da quella dei 15 euro per soli sei mesi di cui state parlando. Forse ieri alla Camera non c'è stata soltanto una sconcertante miscela di irresponsabilità e incapacità. In ogni caso questa tesi, che il Governo stesso sta accreditando nelle ultime ore, è finanche più allarmante. Non è difficile comprendere quanto questo rovinoso capitombolo leda la credibilità stessa del nostro Paese e quanto questo minacci di pesare sulle diverse e delicate trattative in corso con l'Europa, dal PNRR al nuovo Patto di stabilità. L'aumentato nuovo *deficit* di credibilità, per il quale dobbiamo davvero ringraziare il Governo e la maggioranza, rende ancora più ipotetici i saldi del DEF che ci accingiamo a rivotare. Sul fatto che si tratti di un DEF decisamente virtuale credo che ormai ci siano ben pochi dubbi. Bankitalia ha chiarito che gli obiettivi di crescita sono realizzabili soltanto con un'efficace attuazione del PNRR. Ma noi sappiamo - anzi, temiamo - che completare tutti gli obiettivi del Piano sarà impossibile e che a essere sacrificato sarà il provvedimento più caro e comunque molto caro a moltissime famiglie, sul quale peraltro il Governo Conte II giustamente puntò, cioè quello che riguardava gli asili nido. Vi dite preoccupati del calo demografico, vi riempite la bocca di retorica nazionalista, ma poi vi guardate bene dal fare ciò che servirebbe, e cioè raddoppiare l'assegno unico - com'è stato ricordato giustamente anche ieri, e come sarebbe giusto - o mettere a terra i progetti degli asili nido del PNRR. PNRR. Questo non è semplicemente molto grave, non è semplicemente una scelta profondamente sbagliata: dimostra chiaramente come nelle vostre azioni ci siano molta propaganda, ma pochissimi fatti. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato che sono necessarie cospicue risorse di copertura che appaiono difficili da reperire e cita apertamente delle voci la cui assenza nel DEF è invece molto eloquente. Non avete previsto alcunché per i contratti della pubblica amministrazione adeguati all'inflazione e mettete gelidamente nel conto l'impoverimento di milioni di persone, il cui potere di acquisto, eroso anche dall'aumento dei prezzi dell'energia, è già precipitato nell'ultimo anno. Ancora una volta non c'è traccia di una strategia per affrontare i nodi dello sviluppo e della crescita. Non c'è una politica industriale, non ci sono risposte sul tema enorme della transizione ecologica. non siete cambiati: siete gli stessi che minimizzano l'impatto dei cambiamenti climatici, che si oppongono alle misure proposte dall'Europa, ossia il superamento dei motori a benzina, l'efficientamento energetico degli edifici e la decarbonizzazione. della necessaria e inevitabile tassazione degli extra profitti delle società energetiche, che da tempo invano proponiamo, e che peraltro darebbe anche il segno finalmente di una politica fiscale più equa, più giusta e più progressiva. Ma anche su questo versante dimostrate il vostro interesse a tutelare solo quelli che in questi anni di crisi si sono arricchiti e hanno spesso speculato sulla pelle delle persone. Non mettete un euro sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale: andate nella direzione esattamente opposta; tagliate; prevedete una progressiva diminuzione della spesa sanitaria, dimenticando e rinnegando gli impegni assunti quando la pandemia dimostrò drammaticamente le condizioni quali decenni di tagli avevano ridotto la sanità in questo Paese. Ma tanto a pagare saranno i cittadini più deboli, quelli che non possono permettersi le assicurazioni private. Ma, ancora una volta, perché stupirsi? Voi siete quelli dell'autonomia differenziata. Siete quelli della secessione dei ricchi. Siete quelli che spaccano il Paese e aumentano la diseguaglianza sociale. La progressiva cancellazione di ogni scudo contro l'inflazione lascerà indifese vastissime fasce di popolazione, che necessiterebbero invece dell'unica misura indispensabile, al palo da troppi anni, e cioè gli aumenti salariali. *(Applausi)*. La sola novità di questa nuova versione del DEF è l'inserimento del sostegno alle famiglie con figli, misura in sé naturalmente giusta, ma che impatterà proprio su quel minimo cuneo fiscale per i lavoratori previsto dal DEF precedente, e cioè dalla versione che avevamo conosciuto fino a ieri. Per concludere, Presidente, nell'apparente mancanza di visione di questo DEF, c'è in realtà una visione tanto nitida, dal nostro punto di vista, quanto inaccettabile: quella di un Governo che scarica tutti i costi della crisi sui soggetti più deboli, sulle fasce più povere, sulle aziende in maggiore difficoltà, sui lavoratori, finanche e addirittura sui malati. Il nostro progetto quello che abbiamo cominciato a definire nella risoluzione unitaria delle opposizioni - è radicalmente alternativo al vostro, a una visione priva di solidarietà, fondata sulla diseguaglianza, che noi contrastiamo oggi con forza e che con la stessa forza contrasteremo anche domani.

solo una settimana fa in quest'Aula abbiamo assistito a un braccio di ferro tra Governo e maggioranza sugli emendamenti al decreto-legge sull'immigrazione: una sorta di balletto andato oltre il tempo massimo, con una forzatura regolamentare sulla modifica dell'emendamento Gasparri appena poco prima del voto. Ieri mattina, alla Camera, rispondendo a un *question time,* il ministro Casellati ha tenuto a sottolineare che le iniziative di modifica della legge elettorale per i sindaci non hanno il benestare politico dell'Esecutivo. Nel pomeriggio, poi, abbiamo assistito a un fatto di una gravità inaudita, consumatosi mentre il Presidente del Consiglio era in visita ufficiale a Londra e a poche ore dalla partenza del Ministro dell'economia per il vertice Ecofin. Come se non bastasse, questa mattina apprendiamo dai giornali che la modifica della maggioranza alla propria risoluzione sul DEF - relativa alla sanità - è stata apportata all'insaputa del Ministero dell'economia, con i tecnici e gli uomini del Ministro su tutte le furie. Ora, se tre indizi, gravi, precisi e concordanti - come si dice in gergo legale - fanno una prova, la domanda è lecita: cosa sta avvenendo tra i parlamentari della maggioranza e il Governo, tra le forze che sostengono l'Esecutivo? Cose come quelle accadute ieri sera non accadono mai per caso e non possono nemmeno essere rubricate - come ha detto a caldo il ministro Giorgetti - come una mancanza di consapevolezza dei parlamentari. Ci troviamo di fronte a due ipotesi, Presidente, entrambe altamente sconfortanti: la prima è che siamo davanti a uno sfilacciamento della compagine di maggioranza, con i parlamentari che non si sentono abbastanza coinvolti nei processi decisionali e nelle scelte politiche, fino a produrre iniziative autonome e contrarie anche all'indirizzo del Governo. E, se questo accade dopo appena sette mesi dall'inizio della legislatura, saremmo davanti a un fatto molto grave. Non voglio pensare a cosa succederà allora più avanti, quando il centrodestra affronterà un fisiologico calo nei sondaggi; quando prevedibilmente qualche attesa di oggi dei singoli deputati darà vita a dispiaceri; quando bisognerà dimostrare di avere tempra politica. Una coalizione

tra i partiti che sostengono la maggioranza: una crisi che non si può esplicitare agli occhi dell'opinione pubblica, ma che si manifesta con queste modalità sotterranee, con Gruppi parlamentari che producono condizioni di attrito perché i *leader* politici impegnati nella compagine governativa non possono permettersi di darlo a vedere. Qualunque sia la ragione di quanto accaduto ieri, escludendo, per rispetto delle istituzioni, che si sia trattato solo di una tragica inconsapevolezza delle responsabilità del proprio ruolo di parlamentari, non dobbiamo dimenticare che fuori da questi palazzi c'è un Paese che soffre per la perdita di potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, per i mutui che sono schizzati alle stelle, mentre qui c'è una maggioranza che se ne va a spasso, che non viene neppure a votare per mettere 15 euro in più negli stipendi dei lavoratori per sei mesi. C'è - come abbiamo detto ieri - una risoluzione al DEF che è la fotografia della irrealizzabilità delle promesse elettorali con le quali avete vinto le elezioni; un DEF che non contiene alcun riferimento al superamento della legge Fornero, ma solo tagli come quelli alla spesa sanitaria e quelli che avete già fatto sul reddito di cittadinanza, con la sterilizzazione delle accise della benzina e con la sostanziale cancellazione di Opzione donna. La verità, Presidente, è che l'unica strada per unire crescita e tenuta dei conti pubblici si chiama PNRR: un lavoro ferreo, rigoroso per spendere tutte le risorse, a cominciare da quelle delle Regioni del Sud che ne hanno più bisogno. Sul PNRR abbiamo preso atto delle parole del ministro Fitto che in quest'Aula tre giorni fa ha assicurato che le risorse per il Mezzogiorno non verranno ridotte né distolte. Ma, dopo ieri, ci sia consentito

altro - come il collega Foti stamattina alla Camera - ha affermato che la maggioranza non c'è stata per via della riduzione del numero dei parlamentari. Neanche la logica soccorre questo ragionamento, perché ovviamente portare in Aula 201 deputati è più facile che portarne 316, quelli che erano prima. *(Applausi)*. L'unico nostro sentimento, Presidente, è quello di una profonda - e direi anche giustificata - preoccupazione. Governo e maggioranza dicano parole di verità al Paese; dicano se sono in grado di guidarlo in un momento così importante e delicato. Questo sì che sarebbe un atto di responsabilità dopo le numerose irresponsabilità alle quali abbiamo assistito nei giorni scorsi. In conclusione, Presidente, mantenendo ferma la propria preoccupazione, il Gruppo per le Autonomie - come già dichiarato ieri - voterà favorevolmente, con responsabilità e spirito costruttivo, quelle risoluzioni che indicheranno in modo inequivocabile il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione del Paese, di superamento delle disuguaglianze generazionali, territoriali e di genere per realizzare un tessuto economico più competitivo con il superamento - mi auguro finalmente e non più soltanto verbalmente - delle sperequazioni economiche e strutturali.

e la capacità di riconnettersi con la realtà e con il Paese non guasterebbero. Ieri è accaduto un fatto che - a mio modo di vedere - non può essere declassato come incidente di percorso. Certo, c'è la sensazione che

- secondo cui i *quorum* funzionali sono differenti perché il numero dei parlamentari è modificato, che due più due fa cinque. E stiamo parlando di operazioni semplici: addizioni, sottrazioni, divisioni e non dell'equazione di Schrödinger. Sono semplici operazioni. Certo, c'è un'idea un po' superficiale di come stare nelle Aule parlamentari; quell'idea di una destra da cinepanettone, che deve andare in vacanza c'è un ponte che spinge a partire. Anche questo, francamente, dovrebbe indurre a una cautela nelle argomentazioni e nei toni utilizzati oggi. Ma forse c'è anche di più. Forse c'è anche qualcosa di politico nell'incapacità dimostrata ieri voglio provare a comprendere, magari insieme a voi. Magari c'è una crescente insoddisfazione - oserei definirlo un imbarazzo

fatto. Quei voti che sono mancati ieri pesano, e pesano tanto. Pesano perché dimostrano che, probabilmente, nel tira e molla di una maggioranza complessa, che ha vinto le elezioni in modo netto e vi ricorderò poi su cosa le avete vinte - è chiaro che un DEF insufficiente, senza visione, senza prospettiva e senza soluzioni strutturali, comincia a stare stretto. La coperta comincia a essere davvero molto corta. Allora, guardiamo su cosa avete vinto le elezioni. Sono scomparse le velleità della modificazione delle accise sui carburanti. Dentro quel DEF non vi è alcuna riforma delle pensioni. La Fornero è il vostro traguardo. alcuna riforma di carattere fiscale. Non ci sono i soldi: quindi, la *flat tax* e tutte le promesse che avete fatto riposte nel cassetto. Non c'è una soluzione al tema della crisi demografica. Anzi, su tale questione, che dovrebbe essere una delle principali tematiche su cui elaborare una strategia di cambiamento nel nostro Paese, vige il principio della propaganda: propaganda sul tema dell'immigrazione, propaganda per non risolvere le questioni reali. Ma io vi rammento che, se il dato di decrescita delle nascite rimarrà quello di quest'anno, questo Paese non avrà i conti in ordine per far tornare il tema della tutela del sistema sanitario, del sistema pensionistico, del sistema produttivo, del sistema formativo.

il Paese cresceva e con voi il Paese sta fermo, immobile e il debito cresce. E se il debito cresce, diventa difficile far quadrare i conti. Se il debito cresce, dare una soluzione alle politiche migratorie, ai flussi, alle politiche del lavoro, alle politiche fiscali, alle politiche della giustizia, alle politiche demografiche, diventa estremamente complicato. Quindi, tanto meglio essere indecisi su tutto ed evitare di fare scelte che in qualche modo disallineino

Italia - come può accettare lo spettacolo di una posizione del nostro Paese che non assume scelte sul tema del MES *(Applausi)* e che, parallelamente, vuole andare a trattare la riforma del PNRR o la riforma del Patto di stabilità, non avendo a cuore una visione di sistema con l'Europa? Francamente non lo capisco, né in politica né nella logica.

Al ragionevolissimo ministro Fitto vanno tutti i nostri migliori auguri di buon lavoro, perché ce ne vogliono tanti di auguri per sostenere la tesi che quelle risorse che erano state date dall'Europa per far fare un balzo in avanti in termini di investimenti e di crescita nel nostro Paese oggi devono essere riposte nel cassetto, perché il Paese non è in grado di spenderle

Vi ricordo che le proposte che avete avanzato sono in netta contraddizione l'una con l'altra. Mentre Salvini complicava le norme del codice degli appalti, del ministro Fitto provava a semplificare qualcosa: così non si va da nessuna parte. Come pensate di spiegare a un imprenditore che, per realizzare un'opera di alta velocità, deve cambiare quattro volte le regole nel nostro Paese? *(Applausi)*. Come pensate di attrarre un investitore dall'esterno se l'idea di Paese che avete è che ci sono un'opera di serie A e un'opera di serie B, un territorio di serie A e uno di serie B? B? Penso che lo scaricabarile cominci a non funzionare più e che quella quella discussione sul PNRR sia davvero stata la premessa di quello che è accaduto. Quando un Paese si trova nell'incapacità di dare uno sbocco operativo con soluzioni ai problemi reali esistenti; quando un Paese deve addirittura rinunciare a realizzare gli asili perché non ha le soluzioni pronte

Qualche consiglio ve l'abbiamo dato e ve lo ripetiamo. Un'idea di Paese con il Governo Renzi noi ce l'avevamo. Industria 4.0, per acquisire macchinari, per realizzare impianti, per comprare mezzi di trasporto, per rafforzare il sistema digitale e l'innovazione nel nostro Paese, Paese, è una soluzione e ve l'abbiamo riproposta anche nella discussione sul PNRR. Provate ad ascoltare. Provate ad ascoltare il Paese vero, perché in pochissimo tempo il Paese vero l'avete rimosso completamente dalla vostra Evidentemente siete caduti nel tranello di salotti e discussioni fatte tra di voi, che porteranno poco lontano. Credo sia necessario affrontare questa discussione con una serietà e un atteggiamento diversi rispetto a quello che è prevalso alla Camera. Voi sapete che noi abbiamo detto, fin dal primo momento, senza se e senza ma, no a questo DEF, ma avevamo tenuto un atteggiamento di responsabilità sulla questione dello scostamento. È chiaro che i toni, la discussione di ieri, gli accenti utilizzati, l'incapacità di comprendere quello che è accaduto... prego di concludere.

dico alla collega Paita che noi abbiamo vinto le elezioni con i voti degli italiani. *(Applausi)*. Se ne facciano una ragione lei e tutta l'opposizione.

chiaramente in quest'Aula, a tutta l'Assemblea e soprattutto all'opposizione, che quello che è accaduto ieri non ha alcuna valenza politica, non ha inciso in questa maggioranza. *(Applausi)*. La maggioranza è unita e coesa. E lo dimostriamo oggi, lo abbiamo già dimostrato con il voto sul DEF alla Camera e lo dimostreremo - come abbiamo fatto ieri - anche in quest'Aula al Senato.

di tutto il Parlamento, sia da parte della maggioranza che da parte delle opposizioni. Non si ammettono distrazioni su un provvedimento del genere, proprio perché si tratta di un provvedimento importante. La Costituzione ci dice che che il voto è a maggioranza assoluta, non a maggioranza semplice, e quindi necessita di una condivisione della maggioranza con le opposizioni. Questo significa il voto a maggioranza assoluta. Perciò ripeto Perciò ripeto che è grave quanto è accaduto ieri alla Camera, ma è altrettanto grave quanto è successo dopo, con gli applausi dell'opposizione sul non voto della Camera. un atteggiamento di irresponsabilità che vogliamo sottolineare in quest'Aula per quello che è accaduto. Il voto oggi sul DEF è un voto importante, atteso dalle famiglie, dalle imprese e soprattutto dagli italiani.

dicevo - hanno fatto il Parlamento e questa maggioranza a ritornare subito in Aula. Bene oggi l'impegno del Governo e del ministro Giorgetti a venire in audizione sia alla Camera che al Senato. Senato. In questi mesi il Governo in tema di politica economica sta facendo passi da gigante, e lo voglio ricordare ancora una volta. In poco tempo, a solo un mese dall'insediamento, questo Governo si è fatto carico di una manovra finanziaria che non aveva scritto questa maggioranza, ma aveva scritto un altro Governo, e in quella manovra finanziaria abbiamo cominciato a dare delle risposte ai cittadini, agli italiani. Queste cose forse le dimenticate troppo spesso.

con delle incognite che non riusciamo assolutamente a controllare. Nonostante questo, il DEF è un documento realista, che guarda alla realtà del nostro Paese. Nonostante questo, ci sono dei numeri positivi che ancora oggi il ministro dell'economia Giorgetti ci ha confermato in Commissione bilancio. anzi, ci ha detto che tutti gli operatori del settore guardano con fiducia al futuro dell'Italia: questo è un dato importante e lo voglio ricordare. Nel DEF abbiamo una crescita prevista nel 2024 nel 2025 dell'1,5 per cento. Anche la riduzione del debito oggi è importante

3,4 miliardi di euro, che con una scelta politica ben definita la maggioranza ha deciso di destinare al taglio del cuneo fiscale.

altri 8 miliardi di euro al taglio del cuneo fiscale. Ci siamo già impegnati su questo tema e sul taglio delle tasse. Ci sono poi altri 4,5 miliardi di euro nel 2024 da destinare alla riforma fiscale, la riforma delle riforme, che gli italiani aspettano da cinquant'anni nel nostro Paese, per rigenerare e dare risorse alle famiglie e soprattutto alle imprese. *(Applausi)*. Si tratta quindi di un impegno deciso e forte. Come dicevo, c'è anche la riduzione della pressione fiscale, a noi tanto cara,

alla guerra sono seguiti l'inflazione, la crisi di una banca alle porte dell'Italia e il fallimento delle banche americane. Abbiamo avuto poi l'innalzamento dei tassi delle banche centrali. In questo clima quasi da tempesta perfetta, oggi disegniamo il DEF con coraggio e soprattutto con una visione di Paese. Ci auguriamo che uno di questi fattori possa invece ritrovare un dato

abbiamo fatto scelte politiche, soprattutto in tema di riduzione delle tasse. Si tratta di un tema tanto caro a Forza Italia, che è da sempre un baluardo del presidente Silvio Berlusconi e del nostro Gruppo parlamentare. Ecco perché nel DEF seguiamo tre linee in particolare, tre direttrici, o comunque abbiamo tre indirizzi. Innanzi tutto, occorre uscire dalla straordinarietà del momento. Basta con politiche straordinarie: dobbiamo rendere certa tutta una serie di misure per gli italiani e sicuramente anche per le famiglie in difficoltà. Dobbiamo ridurre il *deficit* della pubblica amministrazione rispetto al PIL e poi, soprattutto, dobbiamo

nel Documento di economia e finanza. Cito poi l'utilizzo di tutti i fondi del PNRR. State tranquilli: utilizzeremo bene tutti i fondi,

dopo averlo fatto in Consiglio dei ministri, lo abbiamo fatto ieri in Senato e lo ribadiamo oggi. Questo è un Documento di economia e finanza che getta le basi oggi di un percorso di un percorso di legislatura. Lo voglio dire perché il momento politico più importante della maggioranza, oggi, sarà non soltanto la nostra coesione, ma la visione di legislatura, che è molto importante. *(Applausi)*. Questo Documento getta le basi e traccia il percorso perché per uscire dalla crisi economica

che non affronta i problemi del Paese e hanno deciso di dare un segnale forte al loro Governo? *(Applausi)*. Poi, con un ragionamento forse più malizioso, ho pensato: ma non è che forse c'è un problema all'interno della maggioranza, al cui interno le forze politiche litigano tra loro e qualche componente ha voluto dare un segnale alle altre? E poi, invece, mi sono accorto che, come sempre, la risposta più banale e facile è quella giusta: erano in vacanza, stavano approfittando del ponte.

La cosa più surreale è che, mentre non si va a lavorare quando si deve, si convoca un Consiglio dei ministri il 1° maggio, costringendo tanti lavoratori a lavorare *(Applausi)*, umiliando le forze sociali convocate la sera prima delegittimando totalmente le rappresentanze sociali. Si prevede un provvedimento che è un panno caldo per qualcuno, che però non dà risposte ai temi del precariato e della sicurezza sul lavoro, temi reali, che con la Festa del 1° maggio si cerca sempre di sottolineare al Paese. Questo è doppiamente grave e surreale. Veniamo però alla alla questione del Documento di economia e finanza. Credo sia normale che, quando si fa una campagna elettorale o prima, quando si è opposizione a un Governo, si facciano tante promesse, oppure dall'opposizione si sottolinei come i problemi da risolvere siano facili e che, se quell'opposizione fosse al Governo, avrebbe già risolto tutto. Poi, però, quando si governa è un po' più difficile - devo dire la verità - e lo abbiamo scoperto noi e oggi lo state scoprendo anche però, non siamo di fronte ad alcune parti di un programma elettorale che non vengono attuate, e peraltro avete davanti anche anni per farlo. Qui si tratta di uno sconvolgimento, di uno stravolgimento totale di tutto quello che le forze di maggioranza hanno detto durante la campagna elettorale e che in questo DEF non c'è, o è espresso esattamente al contrario. *(Applausi)* Ricordiamo tutti l'attacco all'austerità dell'Europa fatto negli anni di opposizione e c'è un DEF a crescita zero, un DEF che più austero di così non si può. Ricordiamo tutti la tassa piatta, le pensioni a 1.000 euro, la riforma della legge Fornero, il sostegno all'economia e ai salari e in questo DEF si parla di moderazione salariale? per evitare l'inflazione bisogna fare in modo che le persone siano più povere e non possano spendere? È drammatica questa posizione, espressa chiara e tonda nel DEF. Non parliamo poi della questione degli investimenti e del vostro mondo, il mondo produttivo, quello che sempre ha guardato al centrodestra come modello di riferimento. Voglio tornare sulla questione della Transizione 4.0, avendo letto alcune agenzie di stampa piuttosto surreali. Il piano Industria 4.0, Impresa 4.0 e oggi Transizione 4.0 è stato potenziato nel 2019 con la legge di bilancio e per la prima volta è stato reso triennale, come triennale è la programmazione di bilancio. È per questo che andava rifinanziato dopo tre anni nella legge di bilancio 2022 e non perché c'era la volontà di non finanziarlo, perché da sempre si finanziava con la legge di bilancio, e noi per la prima volta lo abbiamo fatto per tre anni. Che cosa vi hanno fatto di male gli imprenditori per tagliare tutto quello che c'era di buono nelle leggi fatte dal Governo Conte e dai Governi precedenti? *(Applausi)*. È surreale che a farlo siate voi, che avete quel mondo come riferimento culturale. sia del tutto evidente che la totale incoerenza del Governo e della maggioranza cerchi di essere coperta da quelle che si usano chiamare armi di distrazione di massa: alcune *gaffe* certamente ben coordinate e strategiche, le parole usate un po' male e fuori luogo e, dall'altro, tutto il dibattito sul PNRR, che nel DEF viene definito il più grande elemento di sviluppo del Paese, se poi negli interventi in Aula - ricordo il senatore Borghi - e in quelli del Ministro della difesa si dice che non dobbiamo usare tutte le risorse e che dobbiamo tagliare l'utilizzo dei circa 200 miliardi che abbiamo a disposizione per il Paese. Qualcuno dice che la frittata è fatta; altri, come il senatore Damiani, dicono che useremo tutte le risorse. Allora c'è una distrazione totale sui problemi reali del Paese.

poi l'ultima arma di distrazione: i piagnistei con cui si dice che siamo nel momento più difficile; cito il collega Liris, che ieri nel suo intervento ha detto: «È arrivato il Governo Meloni a salvare la Nazione dal precipizio nel quale ci stavate portando». Il presidente Meloni ha detto che state governando nella fase più difficile del Paese e della storia repubblicana. Capisco tutto, ma avrei voluto vedere voi governare il Paese durante la pandemia. Avrei voluto vedere voi governare il Paese in pandemia con voi all'opposizione e con Renzi al Governo.

Questo è il Paese che vi abbiamo lasciato! vi volete occupare di famiglie con figli, ed è sacrosanto. Credo che meriti una discussione approfondita il modo in cui farlo, perché ritengo che la leva fiscale per risolvere il problema della natalità con 13 milioni di italiani che pagano zero d'imposizione fiscale perché stanno al di sotto della *no tax area* sia il modo sbagliato. Quei 13 milioni di italiani hanno certamente figli e non avrebbero alcun beneficio da un taglio delle tasse che già non pagano. Il ministro Giorgetti ha ricordato che bisogna intervenire eliminando le difficoltà e i vincoli che portano le famiglie a non fare figli. Quelle difficoltà sono il precariato, il salario che non c'è o che non è dignitoso. È la direzione opposta a quella verso cui state andando, piuttosto, che ci potrebbe portare a sperare che questo Paese ricominci ad avere un tasso di natalità adeguato.

Ora, però, se questi sono i patrioti, citerei un altro cantante, il maestro Battiato: «Povera patria» (aggiungo: schiacciata dagli abusi di potere)! *(Applausi)*. Colleghi, oggi siamo qui ed è assolutamente legittimo esserci dal punto di vista formale; è legittimo che si ripresenti nelle Aule del Parlamento un Documento modificato dopo che non è stato approvato in un ramo del Parlamento, però c'è un abuso di potere politico. Voi avreste dovuto semplicemente dire che non siete stati capaci di approvare il DEF.

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, innanzi tutto, a nome del Gruppo e, immagino, dell'Assemblea, un abbraccio alla famiglia del collega Augello per questa notizia che ci ha sconvolto.

scusa all'opposizione, che merita rispetto, perché è la maggioranza innanzi tutto che deve garantire i numeri *(Applausi)*, soprattutto sulle leggi di bilancio (ricordiamo che il Parlamento nasce per gestire il bilancio), ma scusa anche ai cittadini che al Governo e al Parlamento chiedono una cosa semplice: che risolvano i problemi, senza polemiche inutili.

Immagino che su questo dovremmo essere d'accordo tutti e vedo che per polemiche inutili ci si divide anche sulle cose elementari. Veniamo al Documento, che è in linea con una legge di bilancio che è stata molto criticata, ma è solida,

costi dell'energia, i tassi d'interesse, la modifica del Patto di stabilità europea, tutti elementi che vanno considerati e valutati. Ci ricordiamo le polemiche sulla legge di bilancio, che a detta dell'opposizione non stanziava misure sufficienti per il costo dell'energia? Ebbene, fortunatamente abbiamo avuto ragione e serviva quello che è servito. Ci ricordiamo i fiumi d'inchiostro versati per la fine degli sconti sui carburanti? Fortunatamente abbiamo fatto così e non abbiamo gettato inutilmente fiumi di risorse pubbliche. non è tutto giusto e perfetto, ma è quello che si può fare in un momento complicato, con prudenza e serietà. Si procede passo dopo passo, aggiornando man mano la programmazione sulla base degli elementi che vengono ad

non necessariamente stanziando risorse. Vi faccio due esempi: la delega fiscale e gli interventi sul mercato del lavoro. La delega fiscale è un intervento che questo Paese aspetta da decenni. L'ultima vera riforma fiscale risale ai primi anni Settanta, figuriamoci. perché è così necessaria questa delega fiscale? Sono tre i punti che fanno capire la necessità di questo intervento di sistema. Funziona il sistema di riscossione? Vi do qualche numero: a fine 2018, il magazzino fiscale, cioè l'ammontare di tasse e imposte non incassate dallo Stato, era pari a 810 miliardi.

Funziona allora il sistema di accertamento? Se una partita IVA o un'impresa fa ricorso e una volta su due vince la partita IVA contro l'Agenzia delle entrate, evidentemente non funziona neanche il sistema di accertamento.

No che non funziona, perché se abbiamo circa l'8 per cento di disoccupazione e solo nel settore turismo e ricezione mancano 300.000 persone, è evidente che qualcosa non funziona nell'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

perché non possiamo permetterci di avere l'8 per cento di disoccupazione, da una parte, e aziende, imprese e artigiani, a cui mancano centinaia di migliaia di lavoratori,

Sì, questo è quello che si vuole fare, però anche in un'ottica in un'ottica di migliore organizzazione del lavoro e della qualità legislativa della produzione del Parlamento. È una buona notizia, colleghi, se si riducono le domande: vuol dire che ci saranno più persone che, anziché chiedere il reddito di cittadinanza, saranno sul mercato del lavoro, che è esattamente quello che prevede la nostra Costituzione. È trascorso da poco il 25 aprile. Quante volte abbiamo sentito dire che la nostra è la Costituzione più bella del mondo? È vero, ma l'abbiamo letta tutta, fino in fondo? L'articolo 2 della nostra al primo comma, dice che abbiamo diritti, ma al secondo dice che abbiamo un dovere inderogabile - espressione molto forte - di solidarietà politica, economica e sociale. È un dovere

primo comma, dice che la Repubblica deve certamente garantire assistenza a chi non ha mezzi di sussistenza, purché sia inabile al lavoro: è semplicissimo. noi abbiamo un grande compito ed un grande onere, garantire i diritti a tutti; i diritti si garantiscono però se ciascuno fa il proprio dovere.

gli studenti dell'Istituto comprensivo «Papa Giovanni XXIII» di Moscufo, in provincia di Pescara, che stanno assistendo ai

Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico si associa alle condoglianze alla famiglia del senatore Augello, al quale ci ha legato un lungo periodo di scontri e anche di battaglie parlamentari, ma sempre molto corretti. Davvero rivolgiamo un abbraccio affettuoso a tutta la sua famiglia. Signor Presidente, la mancata approvazione del DEF, anzi la sua bocciatura, colleghi senatori di maggioranza, è un inedito della storia recente del nostro Parlamento. Questa mattina, con un'affermazione che noi derubrichiamo a ma vorrei essere tranquillizzato dalla maggioranza, il Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si è prima scusato con i propri elettori, fingendo di non ricordare che il Governo della Repubblica serve tutti gli Italiani e che non ci si scusa per gli errori del Governo solo con una parte degli italiani, ma con tutti gli italiani

è uscito il vero volto, quello di una destra che non cambia, signor Presidente, e che contesta le regole, quelle democratiche. Che a nessuno venga in mente, signor Presidente, di toccare le regole di funzionamento della nostra democrazia *(Applausi)*solo perché non ci si trova con i numeri che doverosamente la maggioranza deve garantire. A qualche collega con la memoria limitata ricordo che non è dovuto il voto sullo scostamento di bilancio.

nonostante la voglia di riscriverla, è lì davanti a tutti noi. Il Parlamento è stato unito sullo scostamento di bilancio, per una legge che per fortuna c'è e che rivendichiamo, in momenti eccezionali di emergenza assoluta. Noi oggi non siamo uniti, perché avete un'idea di Paese che noi non condividiamo e ve lo spieghiamo ancora oggi, dopo averlo già fatto ieri (lo hanno fatto con grande chiarezza nel merito del DEF tutti i colleghi del

il ministro Giorgetti è venuto in Commissione ed ha fatto il suo dovere, ma in realtà doveva essere all'Eurogruppo. Spero che vi siate resi conto che, grazie alla vostra incapacità, oggi il Ministro dell'economia, anziché essere lì (se ci è andato, ci è arrivato in ritardo), era qui per tentare di mettere una toppa ad una cosa che si chiama mancanza di senso del funzionamento del Parlamento. Lo diciamo perché da questo buco nero discende quella che consideriamo una totale inadeguatezza a governare.

influenze, malattie o impegni. Quando ci sono assenze, c'è sempre un perché. Noi pensiamo che questa maggioranza non sia adeguata a guidare la settima potenza industriale del pianeta perché non siete ancora riusciti a nutrirvi del senso delle istituzioni, del loro rispetto e del fatto che chi ha responsabilità di Governo non deve occuparsi dei pruriti di una parte rabbiosa dell'elettorato, ma deve servire la bandiera, la Costituzione e il popolo italiano. È solo l'ultimo episodio di scempio di regole non scritte, ma codificate. Nessun Governo finora aveva mostrato in sei mesi tanta sgrammaticatura istituzionale. signor Presidente, è seriamente preoccupato - e lo diciamo con il massimo rispetto - non perché non è al Governo: la bellezza della vita parlamentare è fatta di cicli e questo è il vostro momento, sancito dagli elettori, e ve lo ribadiamo qui noi. Siamo preoccupati perché le notizie rispetto alla nostra scarsa credibilità in Europa ed internazionale si sommano. È di pochi giorni fa la notizia che una nota banca d'affari ha consigliato di uscire dal debito sovrano italiano, che era ed è tuttora più che solido - lo diciamo noi e lo ribadiamo - per orientarsi verso i buoni del tesoro spagnoli.

del tesoro (BTP) nel 2023, a partire da maggio? 178 miliardi. Il costo medio oggi - non so dirvi quale sarà tra qualche mese - è del 3,4 Sfido qualsiasi esponente della maggioranza di Governo a dirci che i prestiti di soli 122 122 miliardi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza siano superiori al costo che ogni mese dobbiamo coprire. *(Applausi)*. E lo copriamo solo se siamo credibili, se siete credibili; ed è questa credibilità che ci preoccupa, signor Presidente. Il problema è proprio questo, la credibilità.

Volete davvero continuare a credere che vi sia un complotto internazionale, che la speculazione mondiale voglia colpire il vostro sacro furore rinnovatore o ancora che vi ribellerete ai *diktat* della *Troika* e a stupidaggini simili? O non volete iniziare a chiedervi se il fatto che l'Italia sia piombata nel buio dello scetticismo e della sfiducia internazionale non sia la diretta conseguenza di questo modo di concepire la vita di governo in Europa e nel mondo? Vi rendete conto che, mentre infuria la crisi internazionale, uno dei membri del G7 si occupa

Dei *rave*? Della protezione speciale dei migranti? Ci occupiamo dello "spacca Italia" di Calderoli? È questa l'idea di Paese nel suo insieme, al tempo della società aperta, sempre più digitale e multietnica? E quali sono la linea e l'indicazione di rotta che arrivano da questo DEF? La linea che arriva da questo DEF non c'è linea, l'ha ricordato il senatore Cottarelli ieri. Non c'è linea nemmeno dentro i numeri reali: un *deficit* tendenziale primario di 8 miliardi, peggiore di quello programmato sei mesi fa, un indebitamento che sale a 10 miliardi nel 2024. Signor Presidente, sono tanti i temi per i quali siamo preoccupati. Si avvii a concludere. le chiedo solo questo - erano lo strumento con cui sarebbero stati coordinati tutti i servizi sanitari offerti sul territorio, soprattutto ai malati cronici. Era prevista la presenza e l'integrazione con i servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili. due anni e mezzo dalla pandemia e dalla crisi più drammatica che abbiamo vissuto, avete detto che li avreste cancellati. Noi non ve lo consentiremo. Signor Presidente, solo un ultimo aspetto. Tutto questo, alla vigilia del 1° maggio. Il 1° maggio, signor Presidente, si manifesta per i diritti dei lavoratori; lo dico e lo ricordo a tutti noi. Scegliete voi qual è la data di riferimento, dal 1° maggio 1886 alla rivoluzione industriale,

Signor Presidente, Governo, colleghi, non posso non esordire con il saluto alla famiglia Augello, per la scomparsa di Andrea persona che, per chi come me viene da questo mondo, è stata da sempre un riferimento per la famiglia del centrodestra e di Fratelli d'Italia e per tutta una scuola politica che non ha mai tradito. *(Applausi)*. Il fatto che la notizia venga resa pubblica durante una seduta del Senato, per me che non credo alle coincidenze, è importante. A lui vada un commosso saluto di ricordo e un abbraccio alla famiglia.

Mi ero ripromesso magari di alzare un po' anche il tono del discorso, ma non sarà così, non soltanto per la scomparsa del collega e amico, ma anche perché

È stato un incidente che non ha avuto e non ha risvolti politici. Chiunque abbia dimestichezza con le tecniche parlamentari e politiche sa bene che i segnali politici vengono dati su provvedimenti minori e non certo sul bilancio, sul DEF e sulla programmazione economico-finanziaria. Sul Documento di economia e finanzia le maggioranze cadono, non si assestano. È evidente che c'è stato un incidente di percorso, ma non per questo è meno grave. chiedo scusa, non certo a voi, non certo ai colleghi che sono dovuti tornare e che fanno parte di una categoria privilegiata, ma chiedo scusa a tutti gli italiani per quello che è accaduto ieri.

ho detto che vi invitavo a scegliere se stare dalla parte dei gufi e degli iettatori o dalla parte di chi tifa Italia. *(Applausi)*. Ho capito da alcuni interventi che voi - o molti di voi - tifate Italia. Spero lo facciate però con convinzione e con atti amministrativi, stando dalla parte della ragione, votando secondo coscienza e non soltanto secondo differenze ideologiche. Un passaggio me lo consentirà il Capogruppo del terzo polo,

ci ha dato una lezione sulle sottrazioni e sulle addizioni, ma tutto mi sarei aspettato tranne che dal terzo polo arrivassero lezioni sulle divisioni. *(Applausi)*. Proprio dal terzo popolo mi sembra abbastanza di cattivo gusto, anche perché non abbiamo mai affondato il coltello nella piaga e sarebbe stato fin troppo semplice. Al collega Boccia, dopo che per dieci anni la sua forza politica è stata al Governo senza aver mai vinto le elezioni, dico che mi sembra grossolano che dia lezioni su come si deve gestire il Paese.

così per quanto riguarda il rapporto *deficit*-PIL: 142 per cento nel 2023, 141 nel 2024, 140 nel 2025.

lapidari e sacri, perché poi consacrano anche chi vince e chi perde le elezioni, ci portano a verificare la previsione di PIL dell'1 per cento nel 2023 e dell'1,5 nel 2024, 800.000 posti di lavoro in più

+2,3 miliardi nel 2024, +2,6 miliardi nel 2025, con un'attenzione nei confronti del territorio e dei dipartimenti di prevenzione per quella ricchezza che essi rappresentano in particolar modo per le aree interne, difficili, montane e marginali e che voi avete impoverito. Ecco la controtendenza. so però chi dobbiamo scomodare per farvi capire che il Governo Meloni sta guidando bene questo Paese. Lo dico perché dopo la CNN, «The Washington Post», la Banca d'Italia, l'Europa e Gentiloni, l'Istat oggi ci dà addirittura la previsione dell'1,8 per cento. Aveva ragione il ministro Giorgetti *(Applausi)* quando diceva che le stime erano fin troppo prudenti. Quando il nostro Presidente del Consiglio a Londra viene accolto con tutti gli onori del caso e ringraziato per quanto sta facendo a capo della nostra Nazione, voi dovete essere soddisfatti, gratificati e orgogliosi proprio perché con questo DEF ci presentiamo ai tavoli europei

anche per quanto riguarda tanti decreti applicativi rispetto alle intenzioni socioeconomiche espresse nel DEF. Oggi in Commissione abbiamo scritto una pagina importante. Questa mattina abbiamo dato abbiamo dato il tempo al ministro Giorgetti di spostarsi dalla Camera al Senato e di arrivare in Commissione bilancio, anche su richiesta dei membri della minoranza.

2023 e più di 4 nel 2024, imputando poi le spese o comunque queste risorse nel 2023 al taglio del cuneo fiscale, all'abbattimento delle aliquote Irpef, alle famiglie, al fattore famiglia e poi, al 2024, per quanto riguarda il decreto fiscale, stiamo operando nella giusta direzione. Ieri ho fatto un riferimento, che vi ha fatto un po' arrabbiare,

È quello che stiamo concedendo. Noi facciamo la politica degli *step*, dei passi e di un moto uniformemente accelerato. Questo ci chiede il nostro Paese e questo l'obiettivo cui stiamo dando seguito. È per questa ragione che, ringraziando il mio Capogruppo, presidente Malan, di aver dato a me la possibilità di fare questa dichiarazione di voto

assoluta dei componenti dell'Assemblea che, mi piace ricordare, per la verità il Senato aveva garantito anche ieri. Pertanto, la votazione

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 1 e 3.

L'ordine del giorno reca: «Votazioni per l'elezione di un componente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e di un componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti». conti». Ricordo che nella seduta di ieri sono stati eletti un componente per ciascuno dei predetti consigli di presidenza, con i nomi indicati dai Gruppi di Non hanno invece avuto la maggioranza assoluta prescritta i candidati Palazzolo e Cardarelli. Anche in questa occasione la votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dal combinato disposto

riceverà una scheda di colore giallo, sulla quale indicherà un solo nominativo. Sarà proclamato eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato.

Signor Presidente, dai giornali di oggi si apprende di una sentenza riguardante alcuni servitori dello Stato. Uno di loro ha così commentato: «Abbiamo combattuto una guerra e ci hanno fatto passare per traditori. Non era così». Sono le parole del generale Subranni, protagonista della fondazione dei ROS, Raggruppamento operativo speciale dell'Arma dei carabinieri. Sono parole che fotografano quanto è avvenuto in Italia: decenni di vergognosi e immotivati processi agli eroi della legalità dell'Arma dei carabinieri, che hanno contrastato la mafia; accuse farneticanti, leggende metropolitane su una trattativa che forse qualcuno vorrebbe ancora alimentare - questa leggenda, una serie continua poi di assoluzioni, che hanno dimostrato che il generale Subranni, il generale Mori, il colonnello De Donno e altri ancora si sono sacrificati per lo Stato e per la legalità, mentre altri hanno alimentato campagne prive di fondamento. Chissà cos'hanno da dire ora, dopo l'ulteriore sentenza della Cassazione, che afferma che chi ha subito ingiuste accuse "non ha commesso il fatto" (questa è la formula). Cos'hanno da dire ad esempio Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia, Roberto Scarpinato e altri, che dovrebbero farsi una domanda e darsi una risposta. Le accuse agli eroi della legalità rappresentano un capitolo di vergogna che non può finire qui. Qualcuno deve pagare per le proprie responsabilità. Sono state distrutte non solo reputazioni, ma anche vite fisiche di persone; a Firenze e altrove qualcuno sta ancora inseguendo fantasmi. Sono lieto anche per l'ulteriore assoluzione che ha riguardato il senatore Marcello Dell'Utri.

per le loro ambigue prestazioni. Sono sempre stato accanto a Subranni, a Mori, a De Donno e a tutti coloro che hanno subito ingiuste accuse, ma le toghe che le hanno alimentate non hanno reso onore alla magistratura, una magistratura che vanta invece eroi come Falcone e Borsellino. Sono vicende che andranno approfondite. Alcuni magistrati che ho citato sono gli stessi che hanno creduto a Scarantino, che si accusava di una orrenda strage. C'è qualcuno che deve spiegare che cosa non ha funzionato. Noi continueremo a cercare la verità, che in alcune procure invece veniva sostituita da teoremi privi di fondamento. La storia non finisce, la storia comincia ora.

Francesco Cardarelli al consiglio di presidenza della Corte dei conti, con una votazione che supera abbondantemente il *quorum* della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, si è conclusa questa procedura